Presidente, onorevoli senatori, signori rappresentanti del Governo, mi sembra opportuno iniziare la mia relazione con una breve premessa storica che dia conto della lunga durata e anche dei ritardi e delle difficoltà con cui il Parlamento italiano ha affrontato il tema della lotta alla mafia. Infatti, la consapevolezza del fenomeno mafioso in sede parlamentare, ai fini della costituzione di una Commissione d'inchiesta, matura soltanto negli anni Sessanta del Novecento. Nella III legislatura si giunse all'istituzione della prima Commissione d'inchiesta, con la legge n. 1720 del 1962. Giungeva così a conclusione dell'*iter* parlamentare un disegno di legge a prima firma del senatore Parri, presentato già nel novembre 1958. Nella relazione introduttiva si trovano esposti più elementi, ritraenti l'evoluzione della mafia, fra cui la precoce sottolineatura che «il problema dell'attività della mafia in Sicilia è divenuto sempre più un problema di importanza nazionale, non soltanto in organi del potere pubblico, ma soprattutto per le sempre più estese e forti correlazioni che il fenomeno ha stabilito con i centri economici e politici della vita nazionale e per i rapporti che ne sono stati accertati in campo internazionale». La legislatura si concluse senza che la Commissione d'inchiesta, appena istituita, avesse dato avvio alle attività. La seconda Commissione parlamentare antimafia fu istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta legge Rognoni-La Torre) sulla scorta dell'emozione suscitata dagli assassinii, il 30 aprile di quell'anno, di Pio La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano e, il 3 settembre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, da poco nominato prefetto di Palermo. Essa non ebbe poteri di inchiesta. Le furono attribuiti i compiti di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa, la conseguente azione dei pubblici poteri e, infine, di suggerire al Parlamento misure legislative e amministrative. Essa terminò i suoi lavori nel 1987, allo scadere della IX legislatura. La terza Commissione parlamentare antimafia fu istituita nella X legislatura, con

dall'offensiva stragista che tolse la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Ciascuna delle successive legislature ha visto approvata una legge istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia. Il testo all'esame dell'Assemblea riproduce pressoché immutato - salvo contenute variazioni di cui adesso darò conto - il testo della legge della legge che istituì la Commissione parlamentare antimafia nella XVI legislatura (legge 4 agosto 2008, n. 132). Le principali variazioni concernono solo alcuni aspetti: aspetti: l'utilizzo della espressione «mafie» al plurale; un aggiornamento dei richiami normativi; una nuova disposizione (articolo 2, comma 1, ultimo periodo), relativa al caso di soppravvenienza, in capo ad un componente della Commissione, delle situazioni previste nella proposta di autoregolamentazione approvata dalla Commissione nella legislatura precedente, da cui discende un obbligo di immediata informazione alla Presidenza della Camera di appartenenza; infine, la previsione che il regolamento interno della Commissione stabilisca il numero massimo dei collaboratori. La legge istitutiva della Commissione antimafia della scorsa legislatura per prima ampliò l'oggetto di analisi alle associazioni straniere, comunque denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. I compiti della Commissione consistono nella verifica, indagine e formulazione di proposte migliorative, su un articolato insieme di temi. Al riguardo, la Commissione riferisce al Parlamento al termine dei lavori, o comunque quando lo ritenga opportuno, in ogni caso a scadenza almeno annuale. I compiti assegnati riprendono l'approfondimento dei seguenti temi e profili: l'attuazione della legge n. 646 del 1982 (la legge «Rognoni-La Torre», che ha introdotto, nel codice penale, l'articolo 416-*bis*, così prevedendo il delitto di associazione di tipo mafioso e che costituisce l'architrave della normativa nonché del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle altre leggi dello Stato e degli indirizzi parlamentari relativi al fenomeno mafioso e alle principali altre organizzazioni criminali; la normativa in materia di collaborazione di giustizia (a questo proposito si nota che il termine entro cui il collaboratore è tenuto a esporre le sue dichiarazioni rimane uno dei profili più controversi della disciplina, che attualmente non prevede possa essere richiesta la proroga, in casi di particolare complessità); l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario agli imputati o condannati per delitto di tipo mafioso, uno strumento decisivo nella lotta contro la criminalità mafiosa; l'azione coordinata di Stato, Regioni ed enti locali, nonché la stipulazione di accordi internazionali in materia di prevenzione delle attività criminali e di cooperazione giudiziaria, anche al fine di creare una spazio giuridico antimafia nell'Unione europea; le trasformazioni del fenomeno mafioso e l'estensione del suo radicamento in Regioni diverse da quelle di insediamento tradizionale; la sua internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni in nuove forme di attività illecite (ad esempio lo sfruttamento di flussi migratori illegali); i connotati socioculturali delle organizzazioni criminali, nelle aree di origine così come in quelle di espansione. Quanto ancora ai rapporti tra mafia e politica, occorre soffermarsi sul fenomeno dell'infiltrazione negli organi amministrativi, con particolare riguardo alla selezione di candidature e gruppi dirigenti e all'incidenza nei successivi momenti storici su delitti e stragi di carattere politico-mafioso. Ancora, vi è il tema della infiltrazione o del condizionamento negli appalti e nelle opere pubbliche, nonché delle forme di accumulazione, investimento e riciclaggio di patrimoni e proventi illeciti, come quello della verifica dell'impatto negativo delle attività mafiose sul sistema produttivo. In ordine alla congruità della normativa antiriciclaggio, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti di impresa, si può osservare che, per quanto riguarda il diritto penale, la fattispecie del reato di riciclaggio è stata progressivamente affinata nel tempo. Tra i profili problematici tuttora dibattuti, vi è quello relativo al fatto che - secondo la legislazione vigente - l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per il reato di riciclaggio. Rimane così sguarnito il cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato che genera l'acquisizione illecita delle disponibilità finanziarie. Secondo più operatori ascoltati dalla Commissione antimafia nel corso della precedente legislatura, ne consegue un'incompiutezza dell'ordito penalistico antiriciclaggio, aspetto che sarà certamente da approfondire. Quanto alla verifica sulla normativa in materia di confisca dei beni e di loro uso sociale e produttivo, si tratta di uno dei nodi problematici, sul piano normativo, soprattutto per quanto attiene alla vendita dei beni immobili definitivamente confiscati. La disciplina vigente è fortemente restrittiva verso la vendita a privati di beni immobili, laddove ammette la vendita a privati di beni aziendali («qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico»). Infine vi è la verifica dell'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, anche consultando le associazioni impegnate nel contrasto alla mafia, nonché il monitoraggio su tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosi negli enti locali e la verifica di efficacia della normativa, inclusa quella circa lo scioglimento degli enti locali e la rimozione degli amministratori. I poteri della Commissione d'inchiesta sono analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, come prevede l'articolo 82 della Costituzione. È però prevista dal disegno di legge una specifica limitazione. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione né limitazioni della libertà personale, a eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni. Per quanto riguarda la struttura della Commissione, è prevista una composizione di 50 membri, come nelle precedenti leggi istitutive. L'articolo 4 del disegno di legge disciplina - mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria - le audizioni a testimonianza. Resta ferma la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Non è di contro opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio. Riguardo poi al segreto di Stato, si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. L'articolo 5 del disegno di legge disciplina la richiesta di atti e di documenti: la Commissione può richiedere copie di atti e documenti agli organi e uffici della pubblica amministrazione, anche di procedimenti giudiziari (oltre che di altre inchieste parlamentari, senza che in tal caso le sia opponibile un segreto funzionale). Degli atti e documenti acquisiti la Commissione stabilisce quali non debbano essere divulgati. L'articolo 6 del disegno di legge prevede il vincolo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto, i collaboratori o chiunque concorra al compimento di atti di inchiesta o ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Il vincolo del segreto è sanzionato penalmente, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Medesima previsione sanzionatoria si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, gli atti e documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione. Infine, la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti. Degli altri quattro disegni di legge in titolo, relativi all'istituzione di una Commissione antimafia nella XVII legislatura, si richiede l'assorbimento. Del loro contenuto, occorre menzionare, per cenni, solo il principale profilo per il quale si abbia significativa variazione rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge n. 93 (d'iniziativa dei senatori Lumia e altri) pone specifica attenzione - entro i compiti della Commissione - all'inchiesta sulle stragi degli anni 1992‑1993. Prevede che, a tal fine, la Commissione possa accedere senza preavviso agli archivi dei Servizi di informazione per la sicurezza. Il disegno di legge n. 656 (d'iniziativa dei senatori De Cristofaro e altri) prevede una riduzione del numero dei componenti della Commissione a 30 membri. Inoltre, prescrive la non opponibilità del segreto di Stato rispetto alla richiesta della Commissione di accesso ad atti in possesso dei Servizi di informazione per la sicurezza dello Stato inerenti a materie di indagine della Commissione. Il disegno di legge n. 722 (d'iniziativa dei senatori Schifani e altri) riproduce, salvo minori variazioni testuali, il dettato della legge istitutiva precedente, la n. 132 del 2008. Infine, il disegno di legge n. 827 (d'iniziativa dei senatori Giarrusso e altri) evidenzia, tra i compiti della Commissione, l'accertamento degli eventi luttuosi del biennio 1992‑1993, con un esplicito riferimento alla presunta trattativa, diretta o indiretta, tra le organizzazioni criminali e apparati, settori o esponenti istituzionali. Anche questo disegno di legge, come il ricordato Atto Senato n. 656, propone di ridurre il numero dei membri della Commissione, prevedendone 40. Esclude, inoltre, la partecipazione di persone condannate per un delitto non colposo, ovvero a pena superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per delitto colposo. Del pari esclude le persone per le quali - per fatti di quella portata - sia stato emesso dall'autorità giudiziaria il decreto che dispone il giudizio o abbia avuto inizio l'azione penale per mezzo della sua promozione da parte del pubblico ministero o sia stato da questi notificato avviso di garanzia. Il disegno di legge, infine, dispone la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato né del segreto d'ufficio né di quello professionale e bancario. Questo è quanto, onorevoli colleghi. Vi ringrazio per l'attenzione e auspico che la Commissione antimafia di questa XVII legislatura possa svolgere al meglio i suoi compiti. È un'aspettativa che non dobbiamo deludere ed è un impegno politico e civile di cui le istituzioni hanno l'obbligo di farsi carico nel supremo interesse della Nazione e della civile convivenza. *(Applausi Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà. [DE Signor Presidente, gentili colleghi, sulle organizzazioni criminali di stampo mafioso in Italia si è detto e si è scritto molto. Dagli anni Sessanta, quando si prese coscienza in sede parlamentare del fenomeno mafioso, fino all'ultima Commissione antimafia della precedente legislatura, sono stati numerosi gli sforzi per investigare e conoscere la malavita nel nostro Paese. L'infiltrazione della criminalità organizzata nel Nord Italia, la penetrazione delle mafie straniere nel nostro Paese, le collaborazioni internazionali tra bande che con il tempo hanno creato dei veri e propri cartelli del crimine - hanno bisogno di un continuo studio e indagine da parte del legislatore e di una sempre maggiore collaborazione con la magistratura e le forze di polizia che quotidianamente si dedicano alla lotta alle mafie. n. 825 istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie, anche straniere. Per la prima volta si parla di «mafie», al plurale. Il fenomeno mafioso infatti non può essere circoscritto alla mafia siciliana o alle altre organizzazioni «tradizionali». Sempre più soggetti stranieri operano nel nostro territorio in maniera trasversale e collaborativa con le associazioni criminali nostrane. Bisogna avere però il coraggio di ammettere che, in alcune occasioni, la lotta alla mafia non è riuscita a centrare completamente l'obiettivo. La memoria va all'inizio della storia repubblicana, quando lo Stato combatté il banditismo pensando in questo modo di sconfiggere la mafia. In quell'epoca cosa nostra era prevalentemente agraria e nemica del nascente sindacalismo contadino in Sicilia, tanto da perpetrare la strage di Portella della Ginestra Nel corso della nostra storia recente sono stati molti i martiri della lotta alla mafia. Vorrei quindi ricordare in questa sede i magistrati, i membri delle forze dell'ordine e anche i politici uccisi nel tentativo di sconfiggere definitivamente il crimine organizzato in Italia. La mafia però sembra essere un passo avanti al legislatore. Quando il Parlamento approva una legge per contrastare uno specifico aspetto del fenomeno mafioso, i criminali hanno già indirizzato la loro attività delinquenziale verso nuovi affari, mutando anche la loro stessa struttura organizzativa. È per questo che tra i poteri d'inchiesta della Commissione penso debba esserci quello di indagare il fenomeno delle ecomafie, ovvero tutte quelle attività illegali delle organizzazioni criminali che arrecano danni all'ambiente. In particolare, sono generalmente definite ecomafie le associazioni criminali dedite al traffico e allo smaltimento illegale di rifiuti e all'abusivismo edilizio su larga scala. Anche attività quali l'escavazione abusiva, il traffico di animali esotici, il saccheggio dei beni archeologici e l'allevamento di animali da combattimento possono essere considerate in questo modo. Quella delle ecomafie è l'unica economia che continua a proliferare anche in un contesto di crisi generale. Un'economia illegale che si regge sull'intreccio tra imprenditori senza scrupoli, politici conniventi, funzionari pubblici infedeli, professionisti senza etica e *boss* criminali. Le mafie ambientali operano la falsificazione di fatture e bilanci, l'evasione fiscale e il riciclaggio, la corruzione, il voto di scambio e la spartizione degli appalti. Semplicemente perché conviene e, tutto sommato, si corrono pochi rischi. Le pene per i reati ambientali, infatti, continuano ad essere quasi limitate alle sanzioni amministrative e l'abbattimento degli edifici continua ad essere una eventualità remota. La fotografia che realizza Legambiente nel suo rapporto annuale sulle ecomafie è implacabile e descrive un Paese dove la criminalità ambientale dilaga e aumenta a dismisura i suoi profitti. Questi i dati relativi al 2012 diffusi da Legambiente nel suo ultimo rapporto sulle ecomafie: 34.120 reati, 28.132 persone denunciate, 161 ordinanze di custodia cautelare, 8.286 sequestri, per un giro di affari di 16,7 miliardi di euro gestito da 302 *clan*, 6 in più rispetto a quelli censiti lo scorso anno. Il 45,7 per cento dei reati è concentrato nelle quattro Regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Sicilia, Calabria e Puglia) seguite dal Lazio, con un numero di reati in crescita rispetto al 2011 (+13,2 Toscana (+15,4 per cento). Prima Regione del Nord Italia, la Liguria. Da segnalare per l'incremento degli illeciti accertati anche la mia Regione, il Veneto, con un +18,9 per cento, e l'Umbria. Crescono anche gli illeciti contro gli animali e la fauna selvatica (+6,4 per cento), sfiorando quota 8.000, a una media di quasi 22 reati al giorno e ha il segno più anche il numero di incendi boschivi che hanno colpito il nostro Paese: esattamente +4,6 È la Campania a guidare anche quest'anno la classifica dell'illegalità ambientale nel nostro Paese, con quasi 5.000 infrazioni accertate, più di 3.000 persone denunciate e 34 arresti. il discorso vale sia per il ciclo illegale del cemento sia per quello dei rifiuti. Proprio in Campania, la pratica criminale di smaltire o riciclare i rifiuti speciali bruciandoli oramai va avanti da molti, troppi anni. Si continua come se niente fosse. Sempre negli stessi luoghi. I reati possono avvenire ogni livello del ciclo dei rifiuti: produzione, trasporto e smaltimento. Il produttore può dichiarare il falso sulla quantità o sulla tipologia di rifiuti da smaltire, oppure incaricare dell'operazione imprese che lavorano sottocosto, essendo a conoscenza del fatto che utilizzeranno metodi illegali. A livello di trasporto, possono venire manomessi i documenti di classificazione della merce, in modo da dirottare il carico o farlo scomparire. Lo sversamento illegale di rifiuti tossici e ordinari, come raccontato dallo scrittore Roberto Saviano in «Gomorra», rappresenta un affare molto lucrativo. Nella «Terra dei Fuochi», quell'area della Campania così conosciuta per i roghi il fatturato dell'ecomafia è stato di 44 miliardi di euro in quattro anni. Un *business* in crescita esponenziale, paragonabile solo all'espansione del mercato della cocaina. Dagli anni Novanta i *clan* camorristici sono i *leader* continentali dello smaltimento dei rifiuti. Il *clan* dei casalesi *in primis*, ma non solo. Anche il *clan* dei Mallardo di Giugliano è molto attivo nella mafia ambientale. L'inquinamento del proprio territorio e il peggioramento della qualità di vita dell'intera comunità, provocando malattie respiratorie, asma, tumori, non sono in grado di fermare l'ansia di enormi profitti immediati da parte dei *clan*. Per abbattere i costi dello smaltimento dei rifiuti, imprenditori senza scrupoli del Nord Italia affidano i loro rifiuti ai *boss* della camorra. Occorre quindi indagare in maniera approfondita i rapporti tra le aziende del Nord e i *clan* che si dedicano allo smaltimento illegale dei rifiuti. Ogni anno centinaia e centinaia di camion portano in Campania vere e proprie montagne di rifiuti che distruggono il territorio e la salute dei cittadini che lì vivono. Come ha scritto Saviano, le campagne del napoletano e del casertano sono «mappamondi della monnezza», riflesso illegale della produzione industriale italiana. Il Sud Italia, quindi, come la discarica abusiva dell'Italia ricca e industrializzata, secondo la triste definizione del vescovo di Nola. L'inquinamento da diossina dei terreni è estremamente pericoloso perché introduce sostanze tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento e raggiunge anche l'uomo. Tutti ci ricordiamo come nel marzo 2008 furono riscontrate presenze di diossina nel latte di bufale provenienti da allevamenti del casertano, attribuite all'inquinamento ambientale. A seguito della notizia, la vendita di prodotti caseari della Campania è diminuita significativamente, non solo in Italia, ma anche all'estero. Il danno provocato dalle mafie ambientali è pertanto molteplice. L'Italia è anche crocevia di traffici internazionali di rifiuti, provenienti dai Paesi europei e destinati in Nigeria, Mozambico, Somalia, Romania e ultimamente anche nei Paesi asiatici. Le ramificazioni delle mafie ambientali si sconfiggono quindi grazie anche ad accordi internazionali. Per questo è fondamentale la creazione di uno spazio giuridico antimafia nell'Unione europea. La criminalità ambientale sa cogliere tutte le nuove opportunità offerte dalla globalizzazione: l'Ufficio centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane segnala che i quantitativi di materiali sequestrati nei nostri porti nel corso del 2012 sono raddoppiati rispetto al 2011, passando da 7.000 a più di 14.000 tonnellate, grazie soprattutto ai cosiddetti cascami, cioè gli scarti riutilizzabili provenienti dalla lavorazione di un altro prodotto. Si tratta di materiali che dovrebbero essere destinati ad alimentare l'economia legale del riciclo e che, invece, finiscono in Corea del Sud (è il caso dei cascami di gomma), in Cina e ad Hong Kong (cascami e avanzi di materie plastiche, destinati al riciclo o alla combustione). Questi flussi garantiscono enormi guadagni ai trafficanti e un doppio danno per l'economia legale: il primo perché si pagano contributi ecologici per attività di trattamento e di riciclo che non vengono effettuate; il secondo perché vengono penalizzate le imprese che operano nella legalità. Consentire alla magistratura e alle forze dell'ordine di intervenire in maniera adeguata, perché frutto di un'attenta ed obiettiva valutazione dei fenomeni criminali, delle loro cause e delle loro conseguenze, dovrebbe essere uno degli obiettivi principali della Commissione parlamentare antimafia. Lottare contro le ecomafie significa quindi tutelare la salute Lottare contro le ecomafie significa quindi tutelare la salute dei cittadini, salvaguardare l'ambiente e il nostro territorio e, da ultimo, incrementare le attività produttive sane del nostro Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle associazioni criminali rappresenta senza dubbio l'espressione di una consapevolezza istituzionale su un fenomeno complesso, nei confronti del quale, oltre agli strumenti normativi e procedurali attualmente vigenti e modificati, abbiamo l'obbligo di fare ancora molto di più. Com'è stato ampiamente evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, la Commissione antimafia rappresenta anche l'espressione di una sorta di emancipazione culturale delle istituzioni rispetto al fenomeno delle mafie, anche perché la sua istituzione parte dagli anni '60. Il lavoro da essa svolto ha rappresentato senza dubbio un valore aggiunto nella lotta alla mafia, sebbene talvolta si sia limitato a semplici posizioni formali. Le mafie rappresentano un *vulnus* economico, culturale, etico e sociale gravissimo per il nostro Paese e il loro contrasto deve essere il primo punto nell'agenda della politica nazionale. Per questo l'istituzione della nuova Commissione parlamentare antimafia rappresenta un passaggio delicato ed essenziale anche in questa legislatura; un passaggio in grado di rinnovare, rimodulando gli strumenti a nostra disposizione, le potenzialità della lotta alla mafia da parte delle istituzioni. Quanto raggiunto alla Camera dei deputati in merito alle proposte di istituzione della Commissione, in uno spirito di trasversalità e di estrema condivisione, deve rappresentare per noi una premessa significativa dalla quale poter partire per rafforzare la volontà politica su un fronte delicato come quello delle politiche e delle iniziative di lotta alla mafia. Mai come in questo momento esse meritano, infatti, una vistosa spinta innovatrice, soprattutto alla luce delle recenti dinamiche connesse alla presunta trattativa tra Stato e cosa nostra, in merito alla quale attendiamo ancora che si faccia chiarezza, e nei confronti della quale l'impulso operativo di una Commissione parlamentare può svolgere senza dubbio un ruolo fondamentale. A vent'anni dalla stagione stragista, le istituzioni non si possono limitare alla retorica o a una entità parlamentare più formale che è realmente operativa: agire e progredire dovrebbero essere le nostre parole d'ordine. Lo scenario entro il quale la mafia e i suoi addentellati si sono evoluti è quello in cui infamia e connivenza si sono mescolati in maniera vergognosa: dinanzi ad esso lo Stato deve agire energicamente in tutti i modi possibili, e soprattutto con tutti gli strumenti possibili. Le proposte di oggi si collocano proprio in quest'ottica, perché consentono al Parlamento di essere protagonista attivo di un percorso di cambiamento, per quanto complesso possa essere. Non voglio peccare di retorica, ma ritengo che proprio con queste basi il Paese possa finalmente fare i conti con la sua storia: una storia recente e oscura che pesa ancora sulla coscienza di tutti gli italiani. a poche ore dalla sentenza per il processo Mori, nell'ambito dell'inchiesta per la trattativa Stato-mafia, tutto questo appare purtroppo ancora più amplificato e significativo. Come ho già avuto modo di evidenziare, a mio parere la nuova Commissione parlamentare antimafia, con un suo rinnovato portato, potrebbe rappresentare un passo in avanti nel percorso di emancipazione culturale, normativa e politica dello Stato nei confronti del fenomeno; un fenomeno in evoluzione e nei confronti del quale dal 1992 sono cominciati a mutare l'approccio e la consapevolezza da parte degli italiani. Nel maggio del 1992, per la prima volta, il Paese ha avuto coscienza della giustizia schiacciata sotto il peso della mafia, e questo ha rappresentato una sorta di iniziazione dell'Italia alla cultura dell'antimafia. La stagione delle stragi, la morte di donne e uomini dello Stato per mano di cosa nostra rappresentano una lente attraverso cui guardare l'evoluzione del nostro Paese. Vent'anni dopo quelle stragi, il nostro Paese è completamente cambiato: oggi c'è un livello di sensibilità e di conoscenza impensabile nei primi anni '90. Nell'opinione pubblica, fino a quel momento, la mafia era additata come qualcosa di astratto lontano dalla realtà e dallo Stato: dopo quegli eventi, la mafia è diventata di colpo qualcosa di reale da combattere. Questa è stata la prima conquista del sacrificio di uomini di Stato; la consapevolezza che la mafia non è solo chi preme un grilletto o sversa nei terreni rifiuti tossici: la mafia è anche chi è connivente e chi ha negoziato con lo Stato permettendo tutto questo. L'infamia maggiore è nella connivenza, nella trattativa tra politica e cosa nostra che, faticosamente e soltanto adesso, sta uscendo allo scoperto. Il Parlamento si deve fare forte di questa consapevolezza, deve valorizzarla e consolidarla, con gli strumenti a disposizione, e veicolarla verso iniziative e proposte che vadano nella direzione di una piena e fattiva lotta alla criminalità. Oggi il Parlamento deve assumersi la responsabilità di migliorare e rafforzare la cultura dell'antimafia che sta prendendo forma in questo Paese. attraverso la costituzione della nuova Commissione antimafia dobbiamo dare voce, con approfondimenti, analisi e confronti, proprio a questa Italia: quella che ha raccolto l'eredità di Falcone e Borsellino; un'Italia di donne e uomini, gente comune e uomini di Stato, senza distinzioni e gerarchie, che sa dire no alla mafia e ai suoi derivati, con orgoglio e con grande dignità. Possiamo farlo soltanto se alla base vi è una volontà politica: quella capace di trasformare le parole in fatti e quella che può invitare tutti alla responsabilità. la volontà politica deve partire dalle piccole azioni e dalle piccole decisioni, dall'applicazione di un codice etico per il Parlamento che possa garantire - a giusta premessa di ogni azione - la trasparenza operativa del singolo. In uno scenario complesso come quello attuale, in cui l'attività dei settori malavitosi risulta essere promiscua e particolarmente invasiva, considerando lo scenario globale entro il quale prende forma, i temi che la Commissione dovrà affrontare sono molteplici. La priorità al momento è quella di mettere in moto il progetto, garantendo oculatezza nella scelta dei componenti, pieno sostegno politico e disponibilità di tutti i Gruppi parlamentari per consentire un celere funzionamento della Commissione già da settembre. La Commissione deve essere chiamata a rispondere su questioni delicate, deve fornire soluzioni e dare indicazioni, non limitarsi ad atti formali. Appare quindi inderogabile il superamento degli steccati e della fumosità della politica in nome di un senso dello Stato e di una responsabilità istituzionale rinnovata, che non può e non deve limitarsi alle parole, ma si deve finalmente tradurre in azioni risolutive per il bene di quell'Italia che vorremmo.

cari cittadini, non è affatto facile rammentare certe affermazioni di taluni amministratori locali in tema di mafia. Ero piccolino, però lo ricordo: un ex sindaco della mia città, negli anni '80, ebbe a dire: «La mafia non esiste». la fece in due situazioni particolari, la prima volta quando a Valderice, una località vicino Trapani,

«La mafia esiste perché ci sono i professionisti dell'antimafia». Lo stesso sindaco negò la cittadinanza onoraria al prefetto Fulvio Sodano. Sempre per questo strano filo conduttore si arriva fino all'attuale sindaco sindaco della mia Trapani, Vito Damiano, che afferma: «Non bisogna parlare di mafia, perché si rischia di dargli soltanto troppa importanza».

i nostri figli devono crescere con una cultura corretta. Si sa che in Italia si preferisce curare piuttosto che prevenire, pertanto si prendono spesso dei provvedimenti solo quando non si può fare altrimenti. Quindi, si è preferito attendere che la mafia avesse già stabilito un sistema organizzativo capillare e che i primi delitti fossero compiuti, vedasi l'offensiva stragista che tolse la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Oggi quel che più preoccupa riguarda gli aspetti inerenti all'ambito funzionale, l'effettivo svolgimento delle funzioni e alla composizione della Commissione antimafia.

e LN-Aut)*. Signor Presidente, senza mancare di rispetto alla Presidenza e a nessuno in quest'Aula, voglio andare oltre qualsiasi tipo di inammissibilità di qualsiasi ordine del giorno, di qualsiasi emendamento Il mio discorso vuole essere quello di una persona normale, di un cittadino normale, di un cittadino senatore della Repubblica normale. È auspicabile, secondo me e secondo noi del Movimento 5 Stelle, incrementare quanto più possibile i poteri e le prerogative attribuite alla Commissione, in modo da rendere più penetranti ed effettivi i controlli e i lavori in genere. emendamenti e i nostri ordini del giorno si muovono. Molta attenzione deve essere prestata all'articolo riguardante la composizione della Commissione antimafia, ove esso non prevede adeguate garanzie, al fine di prevenire risvolti patologici nella nomina dei componenti della Commissione stessa.

nominato la Commissione antimafia inserendo al suo interno dei deputati che sono stati condannati per abuso d'ufficio, per violenza privata; un deputato addirittura, secondo dei rapporti della DIA che parlano chiaro, che parlano chiaro, si dice che abbia rapporti con la famiglia del latitante mafioso Matteo Messina Denaro. E intanto fanno parte di queste Commissioni. Ecco, secondo noi è normale che lì si debba realmente stringere la cinghia. E poiché ‑ ripeto ‑ non posso chiederlo attraverso il Regolamento e non posso farlo in altro modo, chiedo alle forze politiche che sono in quest'Aula di farlo utilizzando il buonsenso. Facciamo in modo che persone rinviate a giudizio o con condanne per reati di mafia non facciano parte della Commissione antimafia della XVII legislatura. Questo ve lo dico io, da cittadino normale: è qualcosa che tutti insieme dobbiamo cercare di andare a spiegare fuori. Voglio prendermi, signor Presidente, insieme a lei insieme a tutti voi, questa responsabilità. Voglio che non ci siano ombre all'interno di questa Commissione.

è opportuno richiamare, brevemente e sinteticamente - come ha già fatto il relatore - la sua evoluzione nel tempo e la sua efficacia. Già con la I Legislatura del 1948 si propose di costituire una Commissione parlamentare d'inchiesta per il problema dell'ordine pubblico in Sicilia. Successivamente, nel 1962, fu istituita la prima Commissione con la legge n.1720. La seconda Commissione parlamentare antimafia fu invece istituita con la legge del 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta legge Rognoni-La Torre); essa, pur non avendo poteri di inchiesta, ebbe attribuiti compiti di verifica per l'attuazione delle leggi antimafia, nonché di accertare la congruità della normativa, l'azione dei pubblici poteri e di indicare al Parlamento misure legislative e amministrative. La terza Commissione, nella X legislatura (con legge n. 94 del 1988), fu dotata di poteri di inchiesta, come le altre che seguiranno. Essa, nelle sue relazioni, dispiegò uno sforzo, sia conoscitivo che propositivo, su come adeguare l'impianto normativo ai cambiamenti intervenuti nella struttura dell'organizzazione mafiosa. Si arrivò alla quarta Commissione nella XI legislatura con il decreto n. 306 del 1992, emanato e convertito in legge in quella fase di emergenza e di offensiva stragista degli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino. Le successive legislature hanno avuto approvata una legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta bicamerale antimafia. Questo breve e sintetico *excursus* della genealogia e dell'evoluzione delle Commissioni parlamentari antimafia si rende necessario per meglio comprendere come sia stato complesso giungere a una realtà che oggi può apparire naturale. Infatti, la Commissione parlamentare antimafia permane ormai come uno strumento giuridico istituzionale imprescindibile per la conoscenza, la lotta e la risoluzione del fenomeno mafioso nel nostro Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, nella XVII legislatura della Repubblica, siamo chiamati a discutere e approvare la legge per l'istituzione della decima Commissione di inchiesta sulla mafia e la criminalità organizzata. Ripercorrendo mentalmente il breve *excursus* appena letto, di cui abbiamo un dettagliato ragguaglio nel *dossier* dell'ufficio studi del Senato, possiamo renderci conto di quanto e come il nostro lavoro quest'oggi sia tutt'altro che un passaggio procedurale obbligato o, addirittura, ripetitivo. ripetitivo. L'istituzione della decima Commissione antimafia infatti rappresenta la riproposizione di uno strumento già consolidato, saggiato nella sua efficacia, ma ancor più da rafforzare, poiché, così come si evolve il fenomeno mafioso, contemporaneamente, anzi anticipandone e troncandone evoluzione e crescita, il nostro lavoro si riveste di volta in volta di maggiore e migliore impegno per una Commissione che deve essere sempre più strumento efficace contro la criminalità organizzata. Da parte nostra, quindi, si rinnova un impegno di elevata responsabilità civica, il dovere di produrre uno strumento straordinario e fondamentale per la vita democratica del Paese e di farlo funzionare bene con un'azione di monitoraggio e controllo del fenomeno mafioso. La struttura delle mafie, la loro azione sul territorio nazionale, i suoi intrecci nella società, con la politica e le istituzioni, in poche parole la sua metamorfosi, rende necessarie continue modifiche alla legge. Oggi la mafia ha cambiato pelle, ma anche DNA, aggiungo io. La mafia con tutte le sue diverse denominazioni regionali e sovraregionali è profondamente incarnata nel corpo sociale ed economico italiano, dedita ad affari illeciti che includono il mercato delle droghe, delle armi, dei rifiuti urbani e tossici e addirittura il mercato degli immigrati clandestini. La criminalità organizzata gode di un miliardario giro di affari mai in crisi. Un enorme illecito, che danneggia paurosamente l'economia nazionale, la spontaneità della creazione di piccole e medie imprese e l'imprenditoria giovanile, specialmente al Sud. Sappiamo bene, però, che il fenomeno coinvolge con modalità diverse anche il Nord del Paese. Dati ed indagini continuamente aggiornati descrivono ormai i territori delle Regioni industrializzate del Settentrione fortemente coinvolte in crescenti affari delle organizzazioni mafiose. Qui, infatti, in tempo di crisi economica, la malavita sta trovando terreno fertile per investire e riciclare enormi somme di denaro di provenienza illecita. Un fenomeno spesso trascurato dalla politica, ma non dagli analisti, riguardo alla sostituzione delle organizzazioni mafiose in prerogative che dovrebbero appartenere allo Stato. Difatti, l'azione dei mafiosi attecchisce meglio laddove la presenza dello Stato è meno presente. Per assenza dello Stato non si deve intendere assenza delle forze dell'ordine: ma penuria e mancanza di servizi, quali scuola, strutture di aggregazione sociale, attività culturali e attività produttive e imprenditoriali. È ormai chiaro che dove lo Stato è assente, dove mancano i servizi e specialmente il lavoro, il crimine mafioso ha gioco facile nell'ingaggiare manovalanza e, spesso, giovani, i quali, non avendo altre prospettive, si lasciano irretire da da criminali senza scrupoli che, sostituendosi allo Stato di diritto, promettono di garantire lavoro, anche se illecito, e protezione. Questo, a mio avviso, è un punto nevralgico della criminalità organizzata su cui la politica dovrebbe concentrare maggiormente i suoi interventi. Tenuto conto dell'evoluzione delle mafie, del loro volume d'affari sempre in crescita, delle loro azioni su scala planetaria attraverso il riciclaggio di ingenti somme di denaro frutto di illeciti in Paesi terzi,

costituisce indubbiamente un significativo strumento di indirizzo e di responsabilità condivise. Ancora una volta, attraverso l'istituzione della Commissione d'inchiesta, siamo chiamati ad approfondire le nostre conoscenze acquisite e ad analizzare l'efficacia degli strumenti istituzionali adottati, migliorandoli laddove necessario. Chiaramente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare tiene certamente conto della conoscenza dei fatti e dei dati qui da me brevemente menzionati e si presenta in linea con le norme che hanno istituito la precedente Commissione, intesa ad estendere l'indagine a tutte le associazioni criminali nazionali e a quelle straniere e di tipo transnazionale che operano nel territorio nazionale. Inoltre, conformemente alle precedenti leggi istitutive, è opportuno conferire alla Commissione il compito di verificare l'attuazione delle leggi adottate contro la criminalità organizzata nelle sue diverse denominazioni, nonché di quelle riguardanti i collaboratori e i testimoni di giustizia e, ancora, quello di accertare la congruità delle leggi relative al regime carcerario previsto per gli imputati o i condannati per delitti di mafia e per il reato di riciclaggio. altro punto fondamentale che la Commissione è chiamata a monitorare riguarda le modalità di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, settore nevralgico per lo sradicamento del *modus operandi* mafioso. Un ulteriore aspetto dell'attività della Commissione d'inchiesta riguarda ancora la verifica dell'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo. La Commissione dovrà, altresì, chiamare tutti i partiti a rinnovare l'adesione al codice di autoregolamentazione, confermando l'impegno a non presentare come candidati alle prossime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, persone soggette a misure cautelari non revocate né annullate, soggetti latitanti o che si trovino in stato di esecuzione detentiva. Più chiaramente, non potranno candidarsi persone inquisite o condannate per associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, traffico illecito di rifiuti. I partiti che non intendano sottoscrivere il suddetto documento di autoregolamentazione dovranno rendere pubbliche motivazioni. Lo stesso testo che approveremo prevede, per i parlamentari, che, in caso di sopravvivenza dopo la costituzione della Commissione di una o più delle succitate circostanze, l'interessato dovrà informare tempestivamente il presidente della Camera di appartenenza. Pertanto, la Commissione dovrà indagare anche sui rapporti tra mafia e politica, poiché purtroppo si tratta di un aspetto sempre attuale della realtà nazionale. L'infiltrazione mafiosa nel sistema economico e produttivo pubblico, laddove sussiste la logica del voto di scambio, è un fenomeno da combattere con vigore sempre maggiore e quindi da interrompere. In tali circostanze bisogna tenere presente che non si garantisce il normale svolgimento della vita democratica italiana, con le ovvie e gravi ripercussioni di ordine sociale, economico e culturale. È ormai chiaro che la mafia trova terreno fertile e prolifera laddove mancano una politica coesa e una struttura sociale culturalmente forte: una società intrisa dei valori e dei principi della giustizia, dell'eguaglianza e della solidarietà è garanzia di autentica libertà in uno Stato di diritto. Dove sono assenti questi valori basilari attecchiscono facilmente la criminalità, la corruzione, il malaffare, ovvero tutti quei mali sociali spesso concatenati fra di Ed è così che si generano quelle dinamiche perverse e pervertenti, che generano anche rapporti di collusione con le amministrazioni pubbliche e che inquinano e indeboliscono le istituzioni e la politica in genere. Ciò sembra accadere in un clima di allarmante indifferenza e assenza critica da parte della stessa società civile, dove la componente etica e morale, più che valore fondante, rischia di ridursi a un *optional,* di cui devono farsi carico solo alcuni: gli eroi occasionali. Concludo questo intervento richiamando tutti a una riflessione etica, al di fuori della quale si rischia di perdere di vista il senso della nostra alta funzione; tale riflessione conduce necessariamente ad una assunzione di responsabilità della Commissione che sarà costituita e del Parlamento, chiamato dai cittadini a fare rispettare e a rafforzare le prerogative e le istanze della vita democratica e dello Stato. In questa situazione, in cui il Paese presenta tale *deficit* etico, si rende ancora più urgente porre l'attenzione alle istanze e alle necessità dei cittadini onesti, laboriosi, dediti al rispetto delle regole, vittime - direttamente o indirettamente - più esposte alle azioni del crimine organizzato. È ormai vitale un cambiamento culturale ancora più forte, una mentalità unita a un'azione che educhi all'etica della responsabilità individuale e sociale. Difatti, la banalizzazione della responsabilità ha finora prodotto enormi guasti alla vita democratica, dove chi ha svolto il proprio dovere con coerenza etica, senza tradire il proprio essere uomo, donna, cittadino, ha pagato (e continua a pagare) anche con la vita. Gente coraggiosa, eroi loro malgrado, che a volte hanno vissuto il dramma di essere lasciati soli da chi, invece, avrebbe dovuto incoraggiarli e proteggerli. Gli esempi sono innumerevoli, dai più eclatanti, quali Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, don Pino Puglisi, Mattarella, Pio La Torre, Livatino, Libero Grassi, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, imprenditori, commercianti e comuni cittadini. La sanità del tessuto sociale dell'Italia va pertanto ristabilita, ma anche rafforzata; all'indispensabile e vitale azione della scuola, della Chiesa, delle associazioni, bisogna quindi affiancare l'etica della responsabilità delle istituzioni e della politica. Il mio è sicuramente anche un appello a tutte le energie sane del Paese, e sono tante, dove al relativismo etico va sostituita - ripeto - l'etica del dovere e della responsabilità, della legalità e della giustizia, per il benessere e il progresso della vita democratica dell'Italia.

sia nella società che in Parlamento, si è discusso sulla necessità o meno di dare vita alla Commissione parlamentare antimafia. Io sono tra quelli che ritengono che la Commissione parlamentare antimafia abbia ancora una funzione, a condizione

in alcuni momenti è stata un faro importante per orientare un Paese dove era prevalente il negazionismo della stessa presenza delle mafie nel nostro territorio, nell'economia e - figurarsi - nella politica. Non basta più,

colleghi, mai il nostro Paese, mai le istituzioni del nostro Paese, mai i Parlamenti che si sono succeduti nella vita dell'Italia, e così i Governi, hanno fatto della lotta alle mafie una prima e grande priorità: mai una priorità intorno a cui raccogliere le migliori energie e la migliore progettualità;

Solo il 13 settembre del 1982 il Parlamento finalmente si svegliò e diede vita a quella legislazione antimafia, il 416-*bis* e l'aggressione ai patrimoni, che sono due pietre miliari, due scelte fondamentali intorno a cui si sono costruite successivamente le migliori scelte della legislazione antimafia. È avvenuto così nei tragici momenti delle stragi del 1992-1993. Falcone aveva un'idea progettuale e sistematica della lotta alle mafie. Quel grande progetto gli fu impedito; la stagione delle stragi di cui oggi molto si discute e quella maledetta trattativa riuscirono a bloccare quella dimensione progettuale. Ecco perché, cari colleghi, oggi siamo chiamati a fare un salto di qualità. Proviamo un po' a sognare ad occhi semiaperti, come diceva un grande intellettuale come Ernst Bloch, e a guardare la nostra società; pensiamo a come la lotta alle mafie potrebbe essere una grande leva in grado di smuovere le montagne dei problemi che abbiamo nel nostro Paese e di dare dinamismo alla nostra economia.

Pensiamo a quanto valore si potrebbe dare alle nuove generazioni recuperando fiducia e speranza nel rapporto con le istituzioni e la politica. Pensiamo a quanta credibilità il nostro Paese potrebbe avere se in Europa riuscisse ad imporre, con un atteggiamento forte e qualificato, uno spazio giuridico antimafia comune, se così riuscisse a fare nel contesto internazionale. È di queste ore la notizia

abbiamo un'opportunità storica e, nei travagli e nelle difficoltà enormi di questa legislatura, un salto di qualità dobbiamo proporlo. Forse la lotta alle mafie potrebbe farci guardare tutti diversamente; forse potrebbe sciogliere dei nodi ancora irrisolti nei rapporti all'interno della maggioranza e con le opposizioni. Insomma, potremmo farla diventare una grande occasione per riformare realmente la politica e per rimuovere gli ostacoli che oggi impediscono alla società italiana di spiccare il volo. La Commissione parlamentare antimafia ha poteri enormi; forse è l'unica realtà istituzionale, tra le democrazie avanzate, che è in grado di intervenire sul potere giudiziario, perché ha gli stessi poteri della magistratura; può intervenire sul potere legislativo, sui Parlamenti, su di noi, perché ha un potere di indirizzo, e sull'Esecutivo. Insomma, ha tutti gli strumenti tutti gli strumenti per guidare questo grande processo di innovazione e cambiamento nella società italiana. Naturalmente dobbiamo crederci. Dobbiamo fare in modo che i parlamentari

Con questo approccio potremmo affrontare la stagione delle stragi del 1992-1993, dire al Paese che, finalmente, le istituzioni, attraverso la Commissione parlamentare antimafia, sono in grado di affrontare quelle terribili verità, preparare il Paese anche alle più profonde e dolorose verità, e fare in modo che quel periodo non sia più un periodo rimosso, che divide, ma un periodo in cui veramente le istituzioni si guardano dentro, capiscono quali siano le responsabilità e si faccia un salto di qualità. È anche un'occasione per allargare la visione della Commissione parlamentare antimafia e giungere ad una visione territoriale aperta.Oggi tutti i territori devono fare i conti con la presenza delle mafie, nessuno escluso. E quando si è negata nel Nord, si è fatto un regalo alle mafie. E quando si è minimizzata nel Nord, si è facilitata la crescita delle mafie e si è arrivati dopo. E anche lì si è organizzata l'antimafia del giorno dopo. Oggi negare e minimizzare è un fatto gravissimo. Dobbiamo invece preparare, organizzare meglio, strutturare una progettualità in grado di colpire le mafie, in tutti i loro aspetti, sul versante militare con una legislazione ancora più avanzata. Pensate se riuscissimo ad approvare delle norme in grado di dire ai *boss* mafiosi: guardate che, qualunque reato voi commettiate, il minimo della pena sarà vent'anni, da vent'anni all'ergastolo! Spezzeremmo il loro meccanismo di *welfare,* di mantenimento delle famiglie, quel riciclo che continuamente sono in grado di attuare perché hanno le risorse per organizzare un *turnover* che le istituzioni democratiche non sono in grado di fare. Bloccheremmo la possibilità a quelli che lasciano il carcere di riprendere l'attività dopo pochi giorni e magari essere colpiti la seconda, la terza volta dalle istituzioni dello Stato con uno spreco di energie e di risorse che oggi non ci possiamo più permettere. in questo Parlamento se riuscissimo a rendere la denuncia obbligatoria per tutte le attività economiche con sanzioni non classicamente di tipo penale, ma di tipo amministrativo, e con incentivi potenti, mai realizzati prima, prima, che vadano nella direzione fiscale e contributiva, per fare di un milione, un milione e mezzo di imprese che oggi pagano il pizzo, dei soggetti di legalità e di sviluppo in grado di dire un no oggettivo, che non dipende più dalla loro volontà contro le mafie! a scelte di questo tipo. Penso sia ormai giunto il tempo di riaprire Pianosa e l'Asinara, di varare tutti insieme una legge sulla incandidabilità di chi è coinvolto in processi di mafia. possibile anche allargare lo spazio d'azione ad altri fenomeni eversivi. Il presidente Grasso più volte ci ha richiamato alla necessità di guardare in modo un po' più profondo a ciò che è avvenuto anche su tale nel Paese. Magari scopriremmo delle connessioni con le organizzazioni mafiose e magari potremmo utilizzare quella metodologia che la storia ha accumulato nella sapienza della Commissione antimafia per fare chiarezza anche lì, su molti fatti che hanno causato lutti, stragi e che hanno compromesso e reso opaca la nostra democrazia. Insomma, colleghi, è una grande occasione, anche in questa legislatura: facciamo in modo che questa legislatura abbia le energie e la forza di compiere questo salto di qualità. La società è pronta, le realtà che operano nella società civile in modo progettuale nel campo dell'antimafia ce lo chiedono. Così noi potremmo indicare finalmente quel salto di qualità

Signor Presidente, colleghi, è ormai consuetudine che tra i primi atti di inizio legislatura vi sia l'approvazione di un provvedimento che ricostituisce l'Antimafia. Ci si muove quindi nel solco della continuità di un impegno che ha portato le Camere ad interrogarsi sia sul fenomeno mafioso nazionale e tradizionale sia - sottolineo in particolare questo profilo - sulle nuove organizzazioni criminali straniere, le quali si sono installate purtroppo sul territorio nazionale parallelamente ai migranti dei rispettivi Paesi d'origine. Non potrebbe essere altrimenti, attesa la gravità della minaccia che lo sviluppo del crimine organizzato rappresenta alla sovranità dello Stato e all'esercizio dei diritti democratici dei cittadini, in Italia come altrove. Il testo che giunge oggi all'esame della nostra Assemblea è il frutto di un lavoro complesso e condiviso, che si conclude sotto il segno dell'unitarietà, come del resto è accaduto a Montecitorio. Vorrei solo sottolineare alcune parti molto rilevanti. L'articolo 1 prevede un mandato di legislatura e un ampio ventaglio di materie di investigazione: dalla gestione dei pentiti all'attuazione del regime carcerario introdotto dall'articolo dalla congruità della legislazione nazionale antimafia allo studio dei mutamenti del fenomeno della criminalità organizzata; dai rapporti tra mafia e politica, con particolare riguardo al condizionamento nella scelta delle persone candidate alle cariche elettive, alle tecniche di difesa nelle gare d'appalto. È importante ancora sottolineare che si indagherà anche sulle associazioni di stampo mafioso straniere, come ho detto prima, in quanto operanti sul territorio italiano, come tra l'altro si fa anche da diverse legislature. importante si rivela l'articolo 2, che riguarda la composizione stessa della Commissione. È prevalsa infatti l'idea di nominare 25 deputati e 25 senatori per renderla ancora più solida e rappresentativa di quanto originariamente previsto.

importante - l'impossibilità di opporre alla Commissione il segreto di Stato rispetto a fatti rientranti nelle sue competenze. Vi è poi una norma che prevede la richiesta di atti e documenti introducendo anche un regime di eccezioni ad un articolo del codice di procedura penale, in modo da permettere l'acquisizione di atti processuali concernenti i procedimenti ancora in corso. quindi la possibilità di deferire ad un regolamento l'organizzazione interna della Commissione. Altro aspetto importante è la procedura accelerata di entrata in vigore, onde agevolare il più possibile la sollecita ricostituzione della Commissione. Come Gruppo della Lega Nord e Autonomie sosterremo certamente l'approvazione del provvedimento che giudichiamo conforme all'interesse di accertare la portata del fenomeno mafioso, vecchio e nuovo, e la congruità delle misure di contrasto adottate per fronteggiarlo. permane il rammarico di constatare come, ad oltre 150 anni dall'unificazione italiana, lo Stato unitario non sia ancora riuscito a venire a capo del problema, che per certi versi si è anche allargato quanto ad aree di insistenza. Desideriamo a questo proposito ricordare che è stata proprio la Lega Nord, in passate legislature, a battersi affinché il campo dell'indagine dell'Antimafia venisse allargato alle Regioni esterne al novero di quelle tradizionalmente infestate dalla grande criminalità organizzata, e non solo per tener conto dell'attività delle triadi cinesi. Cogliamo poi l'occasione per rivendicare ad un Ministro leghista, Roberto Maroni, ora alla testa del nostro movimento, i risultati più egregi in termini di contrasto alle infiltrazioni malavitose. Per questo motivo e perché condividiamo il provvedimento nel suo insieme, preannuncio già che la Lega voterà a favore dell'approvazione della ricostituzione

In passato, con le loro relazioni, le Commissioni hanno dispiegato uno sforzo, oltre che conoscitivo, propositivo su come adeguare l'impianto normativo ai cambiamenti intervenuti nella struttura delle organizzazioni mafiose. e le mafie, Cosa nostra e le altre espressioni della criminalità organizzata, rimangono ancora un problema grave della società italiana e, dunque, della democrazia italiana. Commissione fu istituita e dotata di poteri di inchiesta, nella X legislatura, come poi tutte quelle che l'hanno seguita, le diverse le diverse organizzazioni criminali hanno coltivato vecchi e nuovi traffici, conservando e acquisendo posizioni di potere, soprattutto sul terreno economico, anche attraverso pesanti condizionamenti nella vita politico-istituzionale. della crisi generale che l'economia italiana e quella europea stanno attraversando, con pesanti riflessi negativi anche sulla condizione finanziaria e sulle capacità d'azione dello Stato, la compenetrazione tra criminalità e attività economica è diventata un nodo di estrema rilevanza, specialmente per il Mezzogiorno - lo ha sottolineato il presidente Napolitano l'anno scorso nell'aula *bunker* di Palermo, alla cerimonia di commemorazione del giudice Giovanni Falcone ed è diventata un modo soffocante per ogni possibilità di sviluppo in quelle regioni, in cui la crisi favorisce l'azione predatoria dei *clan* criminali. Questi tendono a porsi come procacciatori di occasioni di lavoro, sia pure irregolari e in nero, in un contesto di disoccupazione crescente e disperata. Il Mezzogiorno rischia di essere stretto in questo nodo scorsoio, in questo circolo vizioso proprio quando l'Italia ha bisogno di un apporto nuovo, delle risorse e delle potenzialità di queste regioni attraverso una loro decisa valorizzazione, in un clima di legalità per aprire la strada di un più intenso, nuovo, diverso e sostenibile sviluppo nazionale. La lotta contro le mafie, dunque, è oggi più che mai una priorità per tutto il Paese. però, dobbiamo proseguire con determinazione e tenacia lungo una strada tracciata e se non sottovalutiamo la persistente gravità della pressione e della minaccia mafiosa, possiamo e dobbiamo anche sentirci più forti che nel passato, proprio per la crescente mobilitazione di coscienze e di energie che si è venuta realizzando nel tempo, per l'eredità morale, per le innovazioni legislative ed ordinamentali sul piano della proiezione internazionale che ci hanno lasciato uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. forti perché l'azione dello Stato, sorretta da un sostegno più largo di opinione anche tra i giovani, ha assestato in questi anni colpi durissimi alla mafia.

una prospettiva di ripresa e di sviluppo economico e sociale, impone uno sforzo di coesione nel senso di un approccio solidale, propositivo, unitario

con una crisi finanziaria acuta, con un palese logoramento del tessuto istituzionale. Per questo noi rimaniamo dell'opinione che garantire stabilità di Governo, mettere in cantiere processi di riforma deve essere anche anche nella fase attuale l'impegno più necessario, più largamente condiviso e sostenuto. Questa è la condizione che può permettere ai giovani - come era nell'auspicio che

ha ricordato che è la lotta di ogni giorno che mostra e prova che l'antimafia è più forte della mafia stessa. C'è parecchio da fare - ha sottolineato il commissario europeo - ma l'attività che ha visto nelle regioni

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo oggi a votare l'ennesima Commissione antimafia. Dobbiamo sicuramente accingerci a questo compito importantissimo facendo una valutazione su ciò che è stata la Commissione antimafia nel nostro Paese. La valutazione sull'operato, le funzioni e i risultati della Commissione antimafia non può che essere fatta di luci e ombre: luci quando la Commissione antimafia ha significato in questo Paese accendere i riflettori in un momento in cui non si parlava di mafia, in cui i rapporti tra la mafia e la politica erano occulti, in cui addirittura la stessa parola mafia non si poteva pronunciare.

colleghi, un compito fondamentale, che non è quello di sostituirci o di sovrapporci all'attività della magistratura, ma quello di utilizzare i nostri poteri per poter capire dove sta andando la mafia prima che essa che essa compia degli atti gravi. La magistratura e le forze dell'ordine intervengono, purtroppo, quando i danni sono già stati compiuti, quando i reati sono già stati commessi, quando ormai è troppo tardi. La possibilità che ci dà una Commissione di inchiesta sulla mafia è di intervenire prima che fatti gravi vengano compiuti. In questo momento, signor Presidente, colleghi, per il Movimento 5 Stelle è fondamentale ed indispensabile accendere i riflettori sulla mafia, in particolare sulla mafia che opera nella finanza. È assolutamente allarmante il dato, che è stato evidenziato anche da altri interventi, la principale attività economico-finanziaria di questo Paese sia divenuto il riciclaggio del denaro delle mafie e della criminalità. È un fatto devastante. Signor Presidente, colleghi, per il Movimento 5 Stelle non è scollegato dal problema delle mafie il fatto che il nostro Paese sia in crisi e sia devastato dalla corruzione, perché sono fenomeni strettamente connessi, che si sostengono a vicenda.

Abbiamo anche il dovere di guardare il nostro presente, che è fatto di un Paese in crisi, in cui le mafie approfittano delle difficoltà economiche per divorare il tessuto delle delle nostre imprese. Le imprese in ginocchio cadono nelle mani della mafia, cadono nelle mani prima dell'usura, poi addirittura delle attività di riciclaggio, e questo purtroppo avviene nella maggior parte delle regioni d'Italia, non più solo nel tessuto economico e industriale del Nord, che ne è devastato. L'Expo è stata oggetto delle attenzioni della mafia, la TAV è sotto indagine per mafia: non c'è una grande opera, non c'è un'attività economica di questo Paese che non cada sotto le grinfie della mafia. della mafia. Dobbiamo domandarci, allora, fino a che punto la mafia è in grado addirittura di paralizzare gli sforzi di qualunque Governo, di qualunque maggioranza per rimettere in piedi l'economia di questo Paese. Se non guardiamo in faccia questo problema, non riusciremo a a fare il servizio che dobbiamo fare per il nostro Paese, per renderlo un Paese migliore. Sicuramente dobbiamo accendere i riflettori anche su un altro aspetto poco indagato della mafia, su cui il Movimento 5 Stelle ha puntato l'attenzione: la mafia, anzi le mafie (perché ormai non sono più solo quelle del nostro Paese) sono diventate un fenomeno geopolitico, operano al pari degli Stati e sono il primo problema per le democrazie occidentali. Questo

Intere Nazioni, anche all'interno dell'Europa, sono cadute in mano alla mafia. Questo è un fatto che noi non possiamo ignorare e per questo avevamo cercato di ampliare - e lo facciamo con i nostri emendamenti - l'oggetto dell'attività di indagine della Commissione.

ma anche di tutte quelle associazioni criminali che hanno colonizzato il nostro Paese. Non ci sfugge che esistono una comunità cinese e una mafia cinese; non ci sfugge che la che la colonizzazione di comunità straniere ha portato ad associazioni di albanesi, di nordafricani o di romeni, che stanno perpetrando in maniera organizzata compiti e fini che vanno a cozzare contro

il fenomeno si sta modernizzando e può interessare anche altre regioni, oltre quelle del Sud. del Sud. La stessa colonizzazione politica di certe regioni sempre occupate dalla stessa coalizione può determinare dei comportamenti similmafiosi. Che differenza c'è

Non esistono associazioni o mafie di serie A o di serie B: sono tutte uguali quelle che obbligano gli imprenditori, in un modo o nell'altro, a pagare

dell'anno scorso, prendeva in considerazione il *project financing* ed evidenziava che forse quello era uno strumento per favorire l'attecchimento di associazioni criminali. Aveva ragione: guarda caso, in molte regioni questo è l'unico strumento che viene utilizzato per bypassare le norme degli appalti pubblici. Questo, secondo il nostro

che il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sia da allargare a tutti

soprattutto in Toscana, in Emilia e in Liguria (le regioni Lombardia e Veneto sono passate in seconda fila: credo che siano già state abbastanza spremute dal punto di vista degli interessi). è necessario valutare anche questo aspetto per non avere il paraocchi e per fare quello che hanno fatto nelle legislature precedenti, perché, come

a dare lustro a questa Commissione e a quello che ha saputo produrre. Noi non faremo mancare il nostro voto con le considerazioni che abbiamo svolto. Riteniamo che chiunque voglia rimandare alla Camera questo provvedimento non faccia l'interesse di questa Commissione, ma quello delle mafie. D'altronde c'è chi dice

antimafia per favorire le associazioni mafiose. il generale Mori è stato assolto. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. È una cosa importante, perché questo Paese deve sapere che i ladri stanno con i ladri e le guardie stanno con le guardie, senza confondere

era accusato di essere colluso con la mafia? Era stato accusato, anche autorevolmente, di non voler contrastare quel fenomeno.

Poi bisogna vedere cosa possiamo fare noi, cosa può fare il Parlamento con la Commissione antimafia per accompagnare questa azione di repressione, naturalmente con leggi, come quelle che ho sempre votato, sul carcere duro e su nessun allentamento della tensione per quanto riguarda la fase repressiva.

e avere danni per decine di milioni di euro, non perché abbia commesso un reato, non perché ci sia stato un fatto specifico, ma perché in fase di prevenzione sociologica, sulla base dei rapporti familiari e di fatti sintomatici, si può arrivare a configurare un pericolo possibile di infiltrazione mafiosa. In soldoni, vogliamo tradurre questo principio? Io parlo il lunedì in ufficio con una persona di origine calabrese, campana o siciliana: quello esce dall'ufficio, va al bar

Presidente, vada a leggersi i rapporti con i quali a Modena, con l'introduzione della *white list*, sono state colpite, con decine di milioni di danni, imprese fatte da modenesi, da gente del luogo stimatissima. I meccanismi sono i seguenti: avete assunto degli operai e dei manovali;

dal prefetto e dal comandante dei carabinieri a dire: sì, non sono stupido, ho visto anch'io che ci sono alcuni nomi che mi ricordo di aver sentito in tribunale, magari chiacchierati. Eccoli: mi potete dire, visto che vogliono iscriversi al

è la fotografia della situazione che abbiamo messo in moto. Per fortuna il Governo ha accolto un ordine del giorno e a fine mese dovrebbero porvi rimedio. Vi riferisco una notizia di

ci sono stati sequestri, corruzione e concussione: lì veramente c'era un collegamento con la 'ndrangheta, dimostrato con un intervento della magistratura, che negli altri casi non c'è stato.

Nord la lotta alla mafia si faccia con questi strumenti, è inevitabile che nessuno assumerà più qualcuno che viene da quelle zone, è inevitabile che nessuno avrà più rapporti con aziende che vengono da quelle zone. Chiedo ai colleghi: le persone oneste che ci sono in Calabria, in Sicilia e in Campania, che non sono malavitose o che hanno sbagliato una volta nella vita, non possono neanche andare a fare i manovali o gli operai? Che devono fare, devono spacciare droga?

di sapere con chi si sta parlando, mentre le istituzioni ti dicono che tu non lo puoi sapere, ma, *a posteriori*, sempre sulla base di queste indagini sociologiche, di parentela e di rapporti di polizia, ti puoi

ma è stato visto aggirarsi un imprenditore calabrese nel loro cantiere. Non ha nessun rapporto con loro, ma si aggirava lì, con nome e cognome. Il titolare della ditta ha ribattuto: se questo è venuto su dopo il terremoto, ha fatto il giro delle sette chiese per trovare lavoro ed è entrato anche nel nostro cantiere, noi che c'entriamo? Bella domanda.

non si sovrapponga alla magistratura, alla polizia e ai carabinieri. Se permettete, non vada neanche riscrivere la storia di ventidue anni fa e delle stragi del 1992 e del 1994, perché forse non è il suo compito. Ci sono cose più urgenti: c'è la mafia di oggi, la camorra di oggi, la 'ndrangheta di oggi e le mafie cinesi di oggi da combattere; e come le combattiamo sul territorio se non studiamo noi mezzi e strumenti efficaci? Su delle questioni di cui ho parlato spero che in quel decreto legge si scriva che, prima di interdire un'azienda, almeno gli indizi siano concordanti, concreti e convergenti, che si dimostri che c'è qualcosa che ha turbato il consiglio di amministrazione, che c'è un elemento di concorrenza che viene leso, che c'è una minaccia, un attentato, un movimento di capitali e non soltanto il fatto che qualcuno è «parente di».

nei confronti di tutti quelli che hanno rapporti con imprese o che assumono persone o hanno collaborazioni con imprese provenienti dal Meridione d'Italia. Ora, io non sono mai stato leghista (e non lo sarò mai perché ho una cultura diversa), ma voi non potete per via indiretta dare ragione alla Lega: Lega: certi atteggiamenti fanno nascere una posizione di contrasto o di diffidenza verso i meridionali che neanche la Lega si sognava di avere. Volevo dire questo, signor Presidente, nella convinzione che tale Commissione davvero saprà affrontare e risolvere efficacemente questi problemi.

si è ricordato in questo dibattito che siamo all'approvazione della sesta legge sulla introduzione della Commissione antimafia. È consapevolezza condivisa e comune che questo non sia un passaggio rituale. Magari fosse possibile non costituire la Commissione antimafia: saremmo arrivati in un'altra Italia! Invece siamo qui, e dobbiamo essere qui come cittadini e come esponenti delle istituzioni! E dobbiamo esserci tutti i giorni, perché la battaglia alle mafie deve essere quotidiana e ininterrotta, condotta con tutti gli strumenti leciti, e deve tradursi in una incessante e instancabile azione da condursi su più fronti. È una battaglia che va condotta con attenzione alle prospettive future, ma anche con attenzione alla prospettiva storica, perché anche la verità sulle stragi di Stato, sui fatti del '91-'92 e, più in generale, sui rapporti tra mafia e politica è importante vorrei dire - non meno importante delle azioni di arresto dei latitanti; non è meno importante di tutte le altre azioni in questo ambito. Bisogna ricostruire anche la storia per debellare questo fenomeno. fenomeno. La battaglia alla mafia deve essere condotta in tutta Italia, contro le mafie italiane, cinesi e russe, con consapevolezza delle infiltrazioni al Nord e al Centro e con la correlata preoccupazione per le distorsioni dei processi economici, delle attività finanziarie e per l'inquinamento dei processi decisionali pubblici. Questa battaglia è una battaglia di civiltà sociale, valoriale, ma anche una battaglia per l'Italia europea. dell'istituzione della Commissione antimafia non deve essere un motivo per sentirsi con la coscienza a posto, ma deve essere un'occasione per riflettere. Non possiamo chiamarci fuori. Non possiamo sentirci solo vittime. Dobbiamo riflettere su ciò che l'inefficienza del sistema ha favorito; su ciò che la crisi economica e sociale e la mancanza di lavoro e di speranza nel futuro per intere generazioni in termini di favoreggiamento di questo fenomeno; su ciò che la perdita di etica e di valori ha determinato, sulla debolezza della politica con la «p» minuscola, sul carico di inefficienze e di di inefficienze e di illegalità che la stessa ha causato. Dobbiamo, quindi, avere la consapevolezza di dover rilanciare la politica con la «P» maiuscola. La lotta alla mafia ha sicuramente bisogno di una politica capace di indipendenza, di autonomia, di scelte coraggiose e forti; di una politica credibile sul piano etico e sul piano della proposta che possa guidare la riscossa del Paese. Ricordiamoci di questo, oggi più che mai; in questo momento così difficile e così incerto. Voglio infine ringraziare, non solo la magistratura e le forze dell'ordine, ma anche «Libera» e tutte le associazioni di volontariato che tutti i giorni testimoniano e combattono le mafie sul campo, a viso aperto e con coraggio. Come non riconoscere in queste testimonianze e in questi esempi il valore della sussidiarietà orizzontale, dell'integrazione tra l'azione dei poteri e la società; la valorizzazione della società stessa, deve essere un compito primario della politica?

***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garavini ed altri, Migliore ed altri, Brunetta ed altri)*

L'ordine del giorno G100 verteva appunto sulla qualità della partecipazione alla Commissione antimafia: possiamo prevedere i migliori strumenti e i migliori ambiti di operatività

è stato vittima di una lupara bianca. Quindi, abbiamo bisogno di orientare l'attività di indagine e del Governo anche all'analisi del fenomeno mafioso nell'ambito complessivo della sua attività geopolitica. Ribadiamo la nostra ferma intenzione di fare luce sulle stragi di mafia e su tutte le stragi rimaste ancora impunite nel nostro Paese e soprattutto riteniamo fondamentale, tanto più in questo momento di gravissima crisi economica, intervenire sui beni ed i patrimoni confiscati ai mafiosi.

metta l'accento, soprattutto per quanto riguarda i delitti di strage, sul biennio 1992-1993. Peraltro, già durante la discussione generale che si è svolta poco fa in questa Aula, abbiamo sentito diversi colleghi senatori intervenuti richiedere un'estensione a 360 gradi, sotto tutti i punti di vista, delle indagini e degli accertamenti dell'istituenda Commissione antimafia.

ci sono invocazioni o richieste che giungono dai familiari delle vittime ma anche dalla società, dai partiti e da rappresentanti istituzionali di altissimo livello affinché si proceda ad accertare fino in fondo le responsabilità personali che in tanti casi non sono state appurate, ma soprattutto a verificare le cause e le responsabilità per cui non si è arrivati a queste individuazioni.

potrebbe, seppur di pochissimo, rallentare i tempi dell'approvazione di questa legge estremamente importante; peraltro la necessità di provvedere a un'individuazione delle responsabilità di stragi e fatti connessi a fenomeni eversivi e mafiosi verificatisi o accaduti in Italia è una necessità vera. Io ricordo che lo stesso primo intervento in Aula da parte proprio di questo Presidente del Senato invocava un ricorso a una Commissione stragi per verificare quello che noi chiediamo. Di fronte a tale prospettazione, non solo del Presidente del Senato ma anche di altri vertici istituzionali, si poneva e si pone una scelta che e cioè l'istituzione di una nuova e autonoma Commissione cosiddetta stragi, oppure l'inserimento all'interno di questo disegno di legge, tra i compiti della Commissione, anche di quello relativo a un'individuazione dei fatti delle stragi e delle responsabilità per la mancata individuazione di questi fenomeni in materia eversiva e mafiosa e, quindi, un inserimento per l'oggetto, così come proponiamo con questo nostro emendamento.

Riteniamo che tale approfondimento e questo tema vadano assegnati alla Commissione oggi istituenda, rendendoci peraltro ben conto dei tempi e del rischio di rallentare l'approvazione del disegno di legge istitutivo della Commissione.

considerato che, in ultima analisi, se tralasciamo un emendamento di questo tipo tralasciamo di approfondire il suo oggetto, in quanto il disegno di legge, così come viene presentato, prospetta essenzialmente di concentrarci sul periodo 1992-1993. Questa è la richiesta. Credo che si possa valutare nell'insieme degli aspetti segnalati.

per tanti aspetti noi stiamo vivendo si estende anche l'attività criminale. In alcuni Stati l'attività criminale mafiosa addirittura è riuscita a introdursi anche nel

dovrebbe riuscire nel tempo ad avere un quadro d'insieme ben definito della situazione criminale organizzata e potrebbe contribuire ad evitare eventuali rimozioni di presidi

che purtroppo in questi anni ha subìto particolari tagli e riduzioni nel personale specializzato e anche nelle retribuzioni a suo tempo previste per il personale che operava in quel settore. chiediamo al Governo di impegnarsi affinché la Direzione investigativa antimafia anche nelle sue sedi distrettuali, sia sempre

oltre al fatto che il rapporto tra politica e criminalità organizzata rappresenta uno degli aspetti più inquietanti. Pertanto, la presenza dello Stato nei territori a rischio è d'obbligo. Per questo riteniamo assurdo quanto disposto da un decreto del Capo della Polizia il 3 giugno 2013 con il quale si è decisa la chiusura del posto fisso operativo di Casapesenna, Comune situato nel territorio dell'Agro aversano, centro e sede dei *clan* malavitosi più pericolosi, dove il suddetto posto di polizia rappresenta per i cittadini l'unico baluardo della legalità presente sul territorio. Una presa di posizione assolutamente doverosa, la nostra, che scaturisce da semplici considerazioni circa la curiosa esigenza, secondo il decreto, di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili in termini di economicità, efficienza ed efficacia. tagli che in buona sostanza, secondo il decreto non andrebbero a minare la capacità operativa della Polizia di Stato sul territorio, che sarebbe garantita dalla vicina presenza della sezione distaccata della squadra mobile di Casal di Principe e del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa. Insomma, un provvedimento che sembra scritto da persone estranee alla storia di un territorio, in cui quel posto fisso, fin dalla sua istituzione nel 1996, ha giocato un ruolo determinante nelle indagini e nelle operazioni che hanno portato alla cattura di capiclan del calibro di Schiavone, Zagaria e Iovine; un provvedimento che sfiora l'assurdo in virtù di opinabilissimi criteri di economicità. Pertanto, chiediamo di impegnare il Governo non solo a revocare immediatamente l'efficacia del decreto di soppressione e a mantenere in vita il posto fisso operativo di Casapesenna, ma anche ad incrementare l'attuale dotazione organica, composta da 24 unità, di cui un solo ispettore, e a stabilizzare il personale che opera, oltretutto in missione, ormai da cinque anni (quindi, con una conseguente riduzione di spesa). Infine, visto che l'unico ipotetico risparmio derivante dalla chiusura di questo posto di polizia sarebbe riconducibile alla locazione dello stabile che ospita gli uffici, si chiede l'impegno a valutare la possibilità di utilizzare quale sede degli stessi uffici uno dei numerosi stabili confiscati ai clan camorristici. Questo permetterebbe di operare nell'ottica del risparmio e della riduzione della spesa, inoltre, tale operazione potrebbe assumere nel territorio dell'Agro aversano un Signor Presidente, con l'ordine del giorno G1.103 proponiamo di impegnare il Governo a revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio della Direzione investigativa antimafia all'aeroporto di Malpensa di Malpensa e a rafforzare l'ufficio, incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, così da garantire un'azione efficace e capillare di contrasto alla criminalità, soprattutto in vista di Expo 2015. A nessuno sfuggirà che gli appalti legati al grande evento sono ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, come sottolineato dalla Direzione nazionale antimafia in una recente relazione e come affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della visita a Milano il 6 maggio scorso. come si motiva allora la chiusura del presidio informativo della DIA collocato presso un aeroporto come quello varesino, che rappresenta il principale crocevia e punto di accesso per per la manifestazione internazionale? L'ubicazione in Malpensa ha una necessità logistico-operativa particolarmente importante per gli scopi investigativi. La soppressione del centro informativo è tanto più incomprensibile se si tiene conto dell'efficienza con la quale il nucleo, istituito il 1° giugno 2000, ha operato in questi anni, offrendo un contributo significativo alle indagini condotte dalla Direzione investigativa antimafia in Lombardia. Le ragioni economiche addotte relativamente alla chiusura risultano inoltre superate dai recenti eventi. Ricordiamo che i locali in uso al nucleo di Malpensa sono stati forniti in concessione dalla SEA SpA ad un costo di 3.500 euro. Il consiglio regionale della Lombardia ha inoltre approvato, il 28 maggio scorso, una mozione nella quale ha manifestato la volontà di compartecipare alla copertura delle spese fisse del presidio. Riteniamo pertanto che in questa fase non sia possibile sopprimere un ufficio fondamentale per garantire la sicurezza collettiva. L'attività del Governo di contrasto alle mafie deve essere potenziata e non diminuita.

il senatore Casson mi fa meglio capire l'intervento del senatore Lumia, anche perché egli ha illustrato con compiutezza, attenzione e professionalità - se di professionalità si può parlare rispetto al mandato parlamentare - le finalità dell'emendamento 1.200.

una parola importantissima, e ricordo che anche il presidente Grasso nel suo discorso d'insediamento in quest'Aula ha fatto riferimento alla necessità che in Italia si chiariscano finalmente le ragioni e le modalità di alcune stragi che, dopo tantissimi anni, sono una pagina oscura della nostra democrazia.

ha tre subordinate e tre congiunzioni. In esso si dice innanzitutto di: «indagare le ragioni per cui non si sono individuate le cause e le responsabilità delle stragi»

troppe congiunzioni e che ci sia rispetto per la compiutezza della lingua italiana. Se lei, senatore Casson, espungesse le due «e», l'emendamento si leggerebbe in questo modo: indagare le ragioni per cui non si sono individuate le cause dei fenomeni mafiosi verificatisi in Italia. A questo punto, l'emendamento sarebbe ultroneo, per la parte che riguarda le cause e le responsabilità dei fenomeni mafiosi verificatisi in Italia. Pertanto, se l'obiettivo è quello di stabilire un collegamento

giorno G1.103 sia assolutamente condivisibile per quanto riguarda il nostro territorio. Capisco che possa esserci la richiesta di una maggiorazione

proprio per il cancro dell'infiltrazione, che si è manifestato e che ha dato obiettivamente, anche per quanto la magistratura può convenirne, risultati positivi per quanto riguarda le indagini e i colpi inferti al fenomeno stesso,

1, lettera *f)*, si legge chiaramente: «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio (...) sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico‑mafioso».

Credo che l'indicazione della lettera *f*), approvata dalla Camera dei deputati, consenta alla Commissione antimafia il più largo ed ampio respiro per poter valutare quanto evidenziato dal presidente Grasso al momento del suo insediamento:

una legge che istituisce la Commissione antimafia: non possiamo, con questa legge, chiedere al Governo, attraverso degli ordini del giorno, di mantenere in vita questo o quell'ufficio di polizia, ancorché, ripeto, le motivazioni possano essere anche condivisibili.

PALMA *(PdL)*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi anche dei miei colleghi di partito e posso anche condividere talune delle perplessità che sono state fin qui espresse. Personalmente, però, con riferimento alla delicatezza della materia oggetto del disegno di legge che stiamo trattando

Del resto è nei fatti che, in più di un'occasione, vi sono stati mancati accertamenti in ordine a vicende di particolare gravità, quali sicuramente sono, senza ombra di dubbio, le stragi ed i fatti connessi a fenomeni eversivi e mafiosi.

mi chiedo se non sia possibile una piccola correzione dell'emendamento stesso, sostanzialmente quando si parla dei «fatti connessi a fenomeni eversivi e mafiosi verificatisi in Italia». Capisco bene qual è il riferimento contenuto nell'emendamento, ma la congiunzione «e», a mio avviso, può aprire la stura anche ad accertamenti che fuoriescono dai fatti squisitamente eversivi mafiosi. Ricordiamo tutti, infatti, che l'aggravante del terrorismo venne contestata con riferimento alle stragi del 1992. credo che l'eliminazione della congiunzione, senza nulla togliere al testo del provvedimento e alla pienezza dei poteri di accertamento della Commissione, si attagli

e per gli effetti che avevano sulla struttura stessa dello Stato, avevano in sé la connotazione tipica dell'eversione e del terrorismo. Dire «fenomeni eversivi e mafiosi» significa consentire anche accertamenti solo sui fenomeni eversivi, che mi sembra nel complesso del testo

Quindi ci saranno molti Comitati che lavoreranno sicuramente sugli obiettivi previsti dalla legge in grado di colpire la mafia di oggi, quella che si è riorganizzata, quella che rappresenta Ci saranno, come sempre è avvenuto nella storia della Commissione antimafia, dei Comitati che indagheranno su quelle vicende che rimangono ancora aperte nella storia recente del nostro Paese. Paese. Preciso per i nostri colleghi che la Commissione parlamentare antimafia utilizza i poteri della magistratura - poteri forti, poteri invasivi naturalmente - non per riprendere un giudicato penale, non per fare il quarto grado di giudizio,

che fu approvato quasi all'unanimità e fu riconosciuto come uno dei momenti più alti della storia e dei lavori della Commissione. Sui problemi eversivi e mafiosi, il presidente Grasso ci ha invitato in questi mesi ad allargare lo sguardo della Commissione, a selezionare quei fenomeni eversivi che possono oggetto d'inchiesta della Commissione parlamentare antimafia perché hanno carattere, appunto, ancora aperto, hanno una funzione e in molti casi si sono toccati con presenze mafiose, e che comunque rimangono oggetto oggetto di un'attenzione più ampia della Commissione, la quale con un Comitato apposito può raggiungere anche quest'altro importante obiettivo, senza necessariamente organizzare una nuova Commissione che, nell'economia del Parlamento e dei nostri lavori, ci porterebbe lontano e non ci aiuterebbe a svolgere bene anche questa attività.

accaduti in Italia». Se questo è lo spirito entro cui si sono mossi i firmatari di questo emendamento, credo che daremmo una risposta al

il punto più delicato di questo emendamento, così come credo anche di quello successivo, l'1.201 (mi correggerà casomai il collega se sbaglio), riguarda proprio questa congiunzione

proprio perché, tra l'altro, a nostro modo di vedere, non si può più parlare di mafia eversiva o non eversiva, in quanto la mafia è eversiva dell'ordinamento costituzionale. L'idea di coloro che hanno proposto questo emendamento è proprio di lasciare questa congiunzione. Sul fatto che l'emendamento possa essere riscritto, secondo l'indicazione del relatore Gotor

aver interpretato bene il senso dell'emendamento e avevo chiesto di fare quella correzione, cioè di togliere la congiunzione «e», proprio per evitare delle confusioni. Prendo atto, alla luce delle dichiarazioni del senatore Casson, che la mia interpretazione era scorretta e che sostanzialmente si intenderebbe, da parte dei presentatori dell'emendamento, far sì che la «Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» si debba interessare di quei fatti squisitamente terroristici ed eversivi che nel passato sono stati oggetto dei lavori della Commissione stragi. E se vado a vedere l'intero testo del disegno di legge istitutivo della Commissione stragi stessa, mi sembra di poter affermare che questo riferimento ai fatti eversivi sia una deviazione rispetto allo schema che regolamenta i lavori della Commissione.

Presidente, per la mia esperienza, ho sempre ritenuto - e lo dico ai colleghi con molta serenità che sullo strumento delle Commissioni d'inchiesta il Parlamento debba procedere con i piedi di piombo. Infatti, ciò che abbiamo constatato nelle passate legislature

non di efficacia, nella ricostruzione storica e politica, con il giusto rigore che si richiede a un legislatore che ha i poteri dell'autorità giudiziaria. Sono stato non solo Presidente della Camera, ma lungamente Vice Presidente della Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi all'epoca dell'approfondimento della vicenda di Ustica, devo dire francamente che l'intervento del senatore Casson un pochino mi preoccupa, perché non c'è un problema di collocazione in questo emiciclo, ma c'è proprio un problema di logica. La Commissione antimafia - come lei credo sappia benissimo, senatore Casson - ha un potere, una rilevanza istituzionale ed un ruolo fondamentale, e credo che tutti noi siamo interessati a salvaguardarlo. Oggi, di fatto, unificare nello stesso organismo la Commissione antimafia e la Commissione stragi (perché a questo molto

dell'ampiezza della materia che si va a toccare. Con quale rischio? Con il rischio che questa Commissione finisca per fare ricostruzioni di carattere storico o altro e si disperda rispetto al necessario approfondimento, che è doveroso, delle materie antimafia, che hanno un'attualità stringente. Sinceramente, se non lo avevo capito bene, dopo l'intervento del senatore Casson l'ho capito benissimo, e rafforzo il giudizio negativo su questo emendamento. Lo dico

delle migliori intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno e in questo modo non stiamo rendendo più efficiente la Commissione antimafia, ma stiamo mettendo in piedi un baraccone che si sa dove inizia e non si sa dove finisce.

*(PD)*. Signor Presidente, ho appena ascoltato l'intervento del presidente Casini e mi rivolgo, con spirito di franchezza e di assoluta colleganza, all'amico e collega Casson. Credo che gli argomenti che il presidente Casini ha portato per avvalorare i suoi suggerimenti siano del tutto condivisibili. Per quali ragioni? Credo che non tanto il senatore Gotor, ma il professor Gotor possa condividere le valutazioni che mi accingo a esporre. Chi ha studiato e si è occupato dei fenomeni stragistici e terroristici che hanno insanguinato drammaticamente il nostro Paese conosce perfettamente le periodizzazioni che caratterizzano la scansione di queste vicende:

Chi si è occupato e ha studiato e scritto su questa materia sa perfettamente che l'intreccio eversivo-mafioso contrassegna la prima metà degli anni Novanta. Peraltro, questa interpretazione, che reputo avvalorata anche da una saggistica e da una bibliografia particolarmente significativa e corposA, è del tutto avvalorata dai responsabili delle associazioni dei familiari delle vittime, i quali insistono per la tipizzazione specifica della natura, delle caratteristiche delle stragi e del terrorismo che ha prodotto lutti lutti così sanguinosi ed immani della storia: pagine non scritte della storia di questo Paese, che certamente meriterebbero di essere riprese e indagate, ma nel rispetto di una distinzione metodologica che diventa a questo punto un criterio di orientamento per districare una materia che va tenuta distinta; altrimenti si rischia una sovrapposizione, che personalmente giudicherei impropria e indebita. Questo, naturalmente, significa che si può trovare una soluzione parlando di «fenomeni eversivi di natura mafiosa».

Se noi vogliamo veramente questa Commissione, se vogliamo veramente una Commissione antimafia, e vogliamo combattere le mafie e le associazioni criminali, dobbiamo, come ha detto il presidente Palma (e mi associo), votare contro questo emendamento. Io invito i colleghi a ritirarlo, perché noi vogliamo la Commissione, vogliamo studiare

Questa grande domanda di verità non deve temere zone d'ombra o possibilità che venga precluso alla Commissione antimafia di indagare. Io vorrei ricordare che ci sono stragi e delitti mafiosi ancora impuniti, sono i più gravi fra i delitti mafiosi, dopo quelli del 1992, ad essere rimasti impuniti: l'uccisione del presidente della Regione siciliana, Mattarella, e quella del capo dell'opposizione. Sono delitti politici collegati ad un quadro eversivo e stragista che va indagato. Noi non dobbiamo avere il timore di accendere la luce su questi gravi fatti che sono accaduti nel nostro Paese. Io penso che non ci sia nessun problema

e fermo restando che la Commissione antimafia suole poi dividersi in Comitati di lavoro, tanto che nella precedente legislatura ce ne furono tredici

e dei fatti connessi a fenomeni di eversione mafiosa accaduti in Italia». Attendo di sapere se i presentatori

Prego, senatore Lumia, poi si rischia di aprire un dibattito infinito, che non è capace di raggiungere il risultato voluto. Si voleva aprire e allargare l'orizzonte della Commissione senza duplicare la Commissione stragi: era possibile farlo attraverso un Comitato, che chiaramente approfondisse alcuni fenomeni eversivi ancora irrisolti nel nostro Paese,

verificare le cause e le responsabilità delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni di eversione mafiosa accaduti in Italia».

Penso che si possa ottenere lo stesso risultato migliorativo con questo punto di sintesi finale

e noi pensiamo che eliminando la congiunzione «e» possa essere raggiunta la soluzione finale produttiva di risultati positivi della Commissione parlamentare antimafia.

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, credo che siamo nella condizione di non dovere neanche chiedere una sospensione per precisare il testo

all'esame dei fenomeni mafiosi e, meglio, di eversione mafiosa. Il fatto che si aggiunga la parola «eversione»

nel momento in cui si esamina, materia squisitamente propria della Commissione parlamentare antimafia per come la competenza viene descritta e limitata dalla lunghissima elencazione di questioni della quale la Commissione stessa dovrà occuparsi.

il Governo lo accetterebbe come raccomandazione, considerato che l'obiettivo che si pone è assolutamente condivisibile, ma bisogna stare attenti ai lo accetterei come raccomandazione se riformulato come invito al Governo a verificare la possibilità di revocare l'efficacia del decreto citato, e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.

Allora, intervengo ora sugli emendamenti suddetti o per dichiarazione di voto? Come preferisce lei, Presidente. Ho bisogno di parlare per un minuto per segnalare un punto al Senato. PRESIDENTE.

sostanzialmente molto poco incisiva rispetto al merito del testo originario, che non è nemmeno una congiunzione, ma una mezza congiunzione in più, noi rinviamo questo testo alla Camera. naturalmente che un'esigenza concreta che c'è nel Paese, cioè quella di far partire la Commissione antimafia rapidamente,

dinanzi a un emendamento che modifica il testo in maniera significativa, per carità, si prendono 15 giorni in più, perché una modifica significativa in qualche modo impone il meccanismo del bicameralismo perfetto nel nostro Paese.

sul complesso degli articoli e poi si può intervenire soltanto per dichiarazione di voto, così come ho chiesto di fare. Diversamente, cosa che il Presidente può fare in termini di Regolamento in quanto può coordinare come meglio crede i lavori dell'Assemblea, è stato fatto un intervento sull'emendamento l'intervento svolto dal presidente Casini mi autorizza a fare un'osservazione di carattere più specificatamente politico sul complesso degli emendamenti, ed anche sugli emendamenti 1.200 e 1.201, che vengono a seguire. Questi

perché, com'è che lei mi suggerisce che non devo parlare degli altri emendamenti? PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento 1.2. FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, faccio un richiamo al Regolamento. Io in sede di dichiarazione di voto posso parlare pure degli Stati Uniti d'America, dell'Australia e del tempo che fa. Lei non mi può dire quello che io devo dire in una dichiarazione di voto. Io in dichiarazione di voto...

hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso». Il contenuto di questo emendamento dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perché è ultroneo, è già compreso nella lettera *f)* dell'articolo 1! Lei, Presidente, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, per dei motivi che sono dei motivi politici, così come precisato dal presidente Casini, noi stiamo votando un emendamento - sul quale non mi sottrarrò al voto, perché mi dichiarerò coerente alla maggioranza - che ritarderà la Commissione antimafia di 15 giorni, se non di più! Domando all'Aula: è più importante allargare il compito che è già previsto, e quindi fare un titolo, oppure mettere in grado la Commissione antimafia di attivarsi immediatamente? *(Applausi

Con l'emendamento originario 1.200 volevamo costituire all'interno della Commissione un Comitato che fosse in grado di intervenire anche sul fenomeno eversivo.

la strage del Rapido 904 ha visto il coinvolgimento anche delle organizzazioni mafiose. Ricorderete tutti la presenza di Pippo Calò, il quale fornì l'esplosivo per quel tipo di strage. noto che intorno a questo argomento vi è divisione ed è vero che quell'emendamento, riformulato, rischia di lasciare la divisione e magari, nell'interpretazione, di precludere alla Commissione, così come formulato nella lettera *f)*, la possibilità di intervenire su fenomeni eversivi con quelle caratteristiche. Siccome l'esperienza parlamentare mi suggerisce che non bisogna essere cocciuti, e ho imparato nella lotta alla mafia che i tempi di maturazione arrivano,

GAL)*. La Commissione parlamentare antimafia poteva addirittura andare avanti e costituirsi anche con quella piccola correzione nelle prossime settimane, con una terza lettura alla Camera, come teorizzato tra l'altro dal presidente Palma. Ma visto che ancora non c'è, noi siamo legati a questa ipotesi, che la maggioranza dell'Aula non ritiene ancora matura. Ma è possibile indagare sulle stragi:

mantenuta e sostenuta, e quindi questa piccola correzione in incidente proposta dal relatore la mettiamo da parte per i futuri lavori della Commissione parlamentare antimafia.

Signor Presidente, a dire la verità, era da parecchio che volevo intervenire, e lo avevo segnalato ripetutamente. Mi rendo però conto che chi si comporta in maniera adeguata, senza alzare i toni, non ha diritto di parlare spesso. Volevo comunque ringraziare il collega Lumia per aver ritirato l'emendamento infatti che questo emendamento, pur sostenendo argomentazioni da considerare, avrebbe rappresentato un elemento di equivoco nell'attività della Commissione, che ha bisogno di approntare nuove sfide e, quindi,

Signor Presidente, all'esito dell'annuncio del senatore Lumia del ritiro dell'emendamento 1.200 avrei potuto fare a meno di intervenire, a dir la verità, sia alcuni passaggi dell'intervento del senatore Lumia sia, principalmente, altri passaggi dell'intervento del senatore Giarrusso, mi impongono di esprimere compiutamente il mio pensiero. allora tutti quanti di uscire fuori da un equivoco. Ha ragione il senatore Ferrara, quando dice che la specificazione di cui agli emendamenti 1.200 e 1.201 era sostanzialmente ultronea rispetto al testo, in quanto quell'attività di valutazione o di verifica delle cause delle stragi o dei fatti connessi all'eversione mafiosa era sostanzialmente ricompresa nei compiti generali già disegnati per la Commissione antimafia e, più specificamente, alla lettera *f Chiunque ha un minimo di dimestichezza con i testi di diritto sa perfettamente che quanto sto affermando corrisponde al vero. Infatti alla lettera *f)*, quando si parla di delitti e stragi di carattere politico-mafioso, non si fa altro che consentire alla Commissione antimafia qualsiasi forma di accertamento in ordine a quei fatti, alle stragi, alle cause, alle ragioni e a quant'altro, e non viene bloccata in questo dall'assenza della parola «eversivo» perché, come tutti quanti noi sappiamo, per le stragi del 1992 è stata contestata la circostanza del terrorismo, con riferimento però ad un fatto intrinsecamente mafioso. Quindi l'emendamento 1.200 non portava acqua al mulino di una maggiore profondità degli accertamenti. Tutt'altro: come in termini più politici di quelli che ho utilizzato e andrò a utilizzare

ha esperienza della Commissione antimafia, sa bene che parlare di un Comitato a cui affidare l'immane lavoro che in tempi pregressi era stato affidato alla Commissione stragi è un non dire. Infatti, quei Comitati, signori senatori, per chi non è stato in Commissione antimafia, sono composti da cinque persone, il che equivale a dire che molto probabilmente in quel Comitato non vi sarebbe una rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari, e che sarebbe affidato ad un Comitato di cinque persone un tema così delicato come quello delle stragi eversive (evidentemente non faccio riferimento alle stragi mafiose eversive), per le quali ripetutamente il Parlamento ha ritenuto che vi fosse necessità di una Commissione vera e propria. Qui, senatore Giarrusso, nessuno, ripeto, nessuno, vuole e se lo lasci dire da me e da tanti altri, a partire dal Presidente del Senato, che hanno dedicato la loro vita al contrasto alla criminalità organizzata e che, per il ricordo di tanti amici caduti, ma per il ricordo della propria cronaca personale, mai acconsentirebbero a una vergogna come quella che lei ha immaginato potesse avvenire attraverso la legge. Noi non siamo abituati a percorrere le strade della demagogia, ma da parte di chi lo è forse sarebbe opportuno, signor Presidente, che vi fosse anche un grande rispetto per quest'Aula e per i senatori. Vede, signor Presidente, poco fa in uno di questi interventi qualcuno ha immaginato che la mafia albergasse qui. Questo è grave, signor Presidente: sono affermazioni generiche che minano fino in fondo le istituzioni e che non portano nessuna acqua al mulino della politica. Queste sono le ragioni per cui noi ringraziamo il senatore Lumia per avere ritirato l'emendamento, consapevole come egli è, per la pregressa esperienza, che a fronte di una diversità di visione in Aula, è opportuno superare in radice quella diversità, se si vuole un lavoro sereno in Commissione. Per le stesse identiche ragioni, noi voteremo contro l'emendamento presentato dal senatore Giarrusso.

è dimenticati però di una parte importante. Ci siamo concentrati su una congiunzione, dimenticando la parte iniziale per la quale è stata richiesta la riformulazione: accertare i motivi per cui non sono stati individuati L'obiettivo di questo emendamento (dell'emendamento che avevamo presentato noi) non è quello di indagare sulle stragi politico-mafiose come previsto dal comma

si sia steso un velo e si sia fatto depistaggio. Era questo l'obiettivo di quell'emendamento, e questo è stato nascosto dietro un dibattito su una congiunzione. Questo era quello che volevo sottolineare. È un argomento divisivo, quando si parla di mafia, Presidente, sono francamente sorpreso ed esterrefatto, per un fatto molto semplice, perché, lo ripeto, è la mia prima esperienza in quest'Aula, e io a quest'Aula porto molto rispetto. allora perché il mondo esterno è completamente distante, di fronte alla facile e sterile demagogia che si fa su un argomento che trovo del tutto indifferente. La domanda iniziale che mi faccio è la seguente: ma se la Commissione di inchiesta sui delitti mafiosi viene istituita, a che cosa serve, se non indaga sulle stragi di mafia?

forse a qualcuno sarà sfuggito, infatti, che c'è stata oggi una sentenza del tribunale di Palermo che ha restituito dignità a degli ufficiali dei Carabinieri che hanno correttamente operato sul territorio. Credo che vada dunque superata la sterile polemica che si è insinuata in quest'Aula e che vada ripristinato l'interesse collettivo, che forse qui è sfuggito completamente dal nostro obiettivo finale.

Giarrusso - al di là di come la si pensi, se sia cioè più giusto avere una Commissione o due Commissioni e dove si fermano i poteri dell'una e dell'altra considerare quelli che hanno dubbi sull'emendamento che lei ha scritto e che in qualche modo pensano che quell'emendamento non sia utile, perché invece, ad esempio, servirebbe una Commissione stragi,

Ci sono storie, tradizioni e vicende politiche di gente che è morta per questo, di sangue che per questo è stato versato, ben prima che esistesse Grillo, il Movimento 5 Stelle e il vostro autorevolissimo parere.

Presidente, vengo da una città, dalla quale viene anche il senatore Giarrusso, dove la parola mafia per decenni non è stata impressa nei caratteri

non venivano accettati perché contenevano la parola mafia. Catania, infatti, doveva essere come l'isola di Delo, nella quale non si nasce e non si muore: la mafia non esisteva, perché questo consentiva ovviamente di fare di Catania la città nella quale il *business* mafioso e la forza nascosta della mafia potessero intrattenere relazioni anche con quei pezzi della città - pezzi imprenditoriali e della politica che determinavano poi ulteriore forza e ricchezza delle organizzazioni mafiose. Quindi, so di cosa sta parlando il senatore Giarrusso, so di cosa stanno parlando i colleghi del Ora capisco per quale motivo finora la discussione si sia svolta esclusivamente sull'allargamento della competenza della Commissione antimafia e invece i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno annesso grande importanza alla prima parte dell'emendamento che io mi permetto di dire essere un po' ambigua, ma forse lo dico da ex magistrato. Infatti, è ovvio che, nell'indagare le ragioni per cui non si sono individuate le cause e le responsabilità delle stragi, se avessimo alcune alcune pericolose tentazioni che si agitassero nella Commissione antimafia, i primi a poter essere messi sul banco degli imputati potrebbero essere i tanti magistrati che con dedizione, impegno, serietà e indipendenza di questo si sono occupati.

volta esistono), che possono aver contribuito a che le stragi venissero progettate, comunque non le hanno intercettate, hanno consentito che accadessero e talvolta hanno anche fatto di peggio. Questo è un sospetto che aleggia, ed è il sospetto sul quale i colleghi del Movimento 5 Stelle oggi insistono mantenendo il loro emendamento. Mi permetto di dire che se i colleghi rileggono con attenzione del comma 1, come altri colleghi hanno fatto prima, del testo che ci stiamo accingendo ad approvare, che peraltro è identico alla formulazione della proposta Lumia, vedranno che è esattamente sulla connessione tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, sia con riferimento all'infiltrazione della mafia

Quindi, siamo assicurati circa il fatto che esista, nella legge istitutiva della Commissione antimafia, il presidio per cui quell'esigenza giusta possa essere interpretata e possa trovare quindi un seguito Mi sono permessa di dirlo in quanto ho molto apprezzato le parole del collega De Cristofaro, ma penso che da questa discussione dobbiamo uscire tutti sicuri, limpidamente sicuri, che stiamo costruendo un ambito di competenza della Commissione antimafia che sia in grado anche di far luce - poi poi la gerarchia la stabiliranno appunto i commissari stessi - sui diversi punti, ma anche su questa questione, che è centrale: quali rapporti tra la mafia e pezzi della politica, degli apparati (di quello che diavolo sarà, se è stato), sono stati corresponsabili di stragi, di episodi di eversione mafiosa che hanno insanguinato questo Paese. Io credo che con questa lettera il pericolo che questo ambito di indagine sfugga alla Commissione sia escluso. proposito andrà accompagnato da una robusta volontà politica. Per quanto riguarda il mio Gruppo, permettetemi di dirlo - non sto parlando come presidente della 1a Commissione, ma come componente del Gruppo del Partito Democratico - di questo non potete dubitare.